link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

credo sia giusto da parte di tutti noi che siamo qui oggi impegnati nei lavori del Senato esprimere, nel giorno della festa delle Forze armate, il ringraziamento e l'apprezzamento del Senato alle Forze armate per il loro impegno...

applausi)* ...in Italia e all'estero nelle missioni internazionali di pace, secondo i principi e i valori della nostra Costituzione. Credo sia anche giusto esprimere in questa giornata particolare la nostra vicinanza alle famiglie dei caduti nelle Forze armate e dei feriti, che oggi vivono - come vi potete rendere conto - una giornata particolare. Dobbiamo far sentire loro che non li dimentichiamo e gli siamo vicini.

davanti al Senato è in corso una manifestazione di avvocati, con tanto di toga, che distribuiscono un volantino intitolato: «No alla controriforma forense».

scorso: «La verità è che molti avvocati non hanno alcuna tutela negli studi di cui sono dipendenti a mille euro al mese. Costoro saranno vessati oltre che da un novello dirigismo anche dalla "continuità professionale", norma pacificamente incostituzionale, laddove stabilisce che un tuo collega e concorrente decida di privarti dell'iscrizione all'albo e del lavoro sulla base di un giudizio discrezionale». Questo teniamolo presente, quando fra pochi minuti affronteremo la questione delle competenze dei consigli dell'ordine. L'articolo «Anche qualora si ritenesse giusto che a dettare un provvedimento al Parlamento fosse una corporazione, non sarebbe accettabile una riforma che rechi solo danni ai cittadini e alle imprese»; io aggiungo «anche a un intero segmento generazionale del ceto forense». Poi prosegue: «Su chi pensate siano scaricati i costi che dovranno essere sostenuti in termini di tempo e di esborsi per conseguire la formazione professionale e le specializzazioni? Che parcella farà l'avvocato cassazionista nel momento in cui potrà dirsi uno tra i pochi abilitati?». Queste domande dobbiamo porcele perché se le pone il Paese; e dobbiamo anche darvi una risposta. Non possiamo lasciare

In ordine all'emendamento 24.200/1, con il quale si propone di sopprimere all'emendamento 24.200 della Commissione l'inciso «in via esclusiva», rilevo

Già Santi Romano insegnava che le istituzioni si autoproclamano, si automanifestano e quindi si legittimano. Facciamo un esempio: chi ha la rappresentanza dei lavoratori in Italia? L'hanno, congiuntamente e separatamente, le organizzazioni sindacali: la CGIL è rappresentante istituzionale dei lavoratori, la CISL è rappresentante istituzionale dei lavoratori, e lo stesso la UIL. La notazione del collega Li Gotti avrebbe qualche senso se non fossimo in presenza di

per evitare che forti rappresentanze locali possano supplire o tentare di supplire a quella dei consigli dell'ordine. il modello di organizzazione professionale in cui la rappresentanza di una categoria è riservata in via esclusiva a un ente pubblico è quello proprio proprio dell'ordinamento corporativo, che è stato abrogato con un decreto luogotenenziale del 1944

l'ordine dovrebbe rappresentare l'interesse dell'amministrazione della giustizia e della collettività a un corretto esercizio delle funzioni dell'avvocatura. Questo, evidentemente, è molto diverso dalla rappresentanza degli interessi economici e professionali dell'avvocatura. Comunque, almeno eliminiamo l'inciso «in via esclusiva», perché esso implica che nessun altro (nessun sindacato forense, nessuna associazione di avvocati)

76 anni di distanza dalla precedente legge forense.

Sono state proposte soluzioni alternative, che sono state trovate, ma non sono state accettate dall'avvocatura. Se per legge si deve comprimere una categoria rispetto a un'altra,

che si riflette sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Una riflessione è stata sollecitata dal Presidente della Corte di cassazione, che immagino non stia mentendo perché ha fatto pervenire molti documenti scritti

Questo emendamento mira a introdurre nella legge un comma secondo in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del Consiglio dell'ordine, «sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge»

dannosa per lo stesso Consiglio dell'ordine. Se per caso domani ci fosse l'opportunità di chiudere quei locali e aprirne degli altri a un piano diverso non lo si potrà fare perché devono essere i medesimi locali e spazi occupati

Vi rendete conto dell'assurdità di inserire in una legge dello Stato, e una legge di questa importanza, una disposizione che andrebbe riservata al capo ufficio, neanche al Consiglio dell'ordine nazionale? Credo che siamo ancora in tempo per evitare questa mostruosità. Vediamo di prenderci i pochi minuti necessari per ripensarci.

Ma non mi pare che ci siano proposte emendative in tal senso.. E dato che vi è una legge dello Stato che risale ad alcune decine di anni fa ...

di questa legge, il Consiglio dell'ordine di Roma ha sempre avuto allocazione presso la Cassazione. Negli ultimi anni, per motivi logistici, era nata una controversia tra la presidenza della Corte di cassazione e l'Ordine degli avvocati. In questo modo si cercava di risolvere il problema all'allocazione, già contenuta in una legge dello Stato, che nessuno ha chiesto di abrogare. Qui viene esclusivamente regolamentata meglio.

si potrebbe proporre un subemendamento, se fossero d'accordo i colleghi: e cioè che tale ufficio debba essere collocato nel quartiere Prati o nel quartiere Mazzini di Roma. In questo senso si offrirebbe un contributo a quella linearità normativa cui anche il collega Li Gotti si richiamava. Non so se nel dibattito che stiamo svolgendo, calati in una nube della quale siamo prigionieri, si abbia la consapevolezza di ciò che può essere recepito fuori dall'Aula del Senato, signor Presidente. Credo che l'attività normativa dovrebbe portare ad abolire queste previsioni, non certamente a dettagliarle. Il Parlamento esamina dei regolamenti di ordinamento della professione forense, spacciandoli per un'importante riforma: credo che questa norma, che è stata giustamente messa in rilievo dal collega Ichino, sia beffarda rispetto alla richiesta, che viene proposta quotidianamente, di avere una legislazione più semplice e snella, che distingua i grandi compiti del legislatore da quelli delle amministrazioni. Altrimenti si presenti una norma simile a un regolamento di condominio e si indichi pure in quale quartiere di Roma deve essere stabilita la sede dell'avvocatura.

che fa rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Vi è una sentenza passata in giudicato, che, piaccia o non piaccia, è una sentenza passata in giudicato di sfratto. Si tenta ora, con questo emendamento, di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

per un verso con una certa sicumera, per altro in maniera quasi caricaturale e ingiustificata. Così come sono ingiustificate e inopportune le punzecchiature ai colleghi della Lega sul centralismo e sul federalismo: non c'entra proprio niente.

chi è che si investe della causa della parità dei diritti e delle funzioni dei territori e delle rappresentanze e vedremo se sarete coerenti voi. INCOSTANTE

da questo palazzo storico, che in qualche modo simboleggia la presenza unitaria di tutta l'avvocatura italiana nell'ambito del massimo palazzo di giustizia. D'altra parte, si pongono obiettivamente esigenze funzionali,

tutti gli altri ordini. Vi sono, quindi, ragioni che storicamente hanno portato ad individuare la sede dell'ordine forense romano nel massimo palazzo di giustizia italiano. Il fatto che si voglia, attraverso

è una legge ordinaria. Se poi un domani ci saranno esigenze profondamente diverse che comporteranno una modificazione parallela di quella e di questa legge, ciò si potrà fare in futuro, ma oggi le esigenze sono diverse

una sede che dovrebbe essere prevista per legge; trovo tutto questo altissimamente ridicolo. Voglio anche far osservare a chi sta sostenendo queste tesi

siccome abbiamo riportato al Ministro della giustizia, che li stabilisce con decreto, la maggior parte dei provvedimenti più significativi,

con decreto del Ministro della giustizia adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, naturalmente sentendo i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Consiglio nazionale forense, oltre che lo stesso Consiglio nazionale forense. forense. Diversamente, l'asimmetria che si sta sviluppando in questa legge, in cui alcune normative vengono lasciate al Consiglio nazionale forense (che viene a incidere fortemente nella vita dell'avvocatura italiana, condizionando, come hanno scritto i giovani avvocati, la possibilità di sviluppo dell'esercizio di una libera professione) altre norme sono rimesse al Ministro della giustizia, creerà una grandissima confusione. Come ho evidenziato in uno degli interventi precedenti, l'Aula darà vita a una legge che non avrà nessuna caratteristica di organicità

attribuendo alcuni poteri al Ministro della giustizia, altri al Consiglio nazionale forense senza che ci sia ragionevolezza in tali decisioni. Per questo chiedo che l'emendamento 24.203/1 venga accolto.

capisco che spesso il dibattito su un testo così articolato e complesso diventi a sua volta in parte frammentario, in parte farraginoso. Volevo però segnalare che l'emendamento 24.203 della Commissione,

in oggetto. Quindi, è un problema che in realtà è già stato affrontato e superato dalla Commissione.

spiegare le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo. Vorrei aggiungere, tra l'altro, che con l'emendamento proposto dal PD prevediamo che siano sentiti i Consigli degli Ordini territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense

che esprimeremo su questo articolo è motivato non solo dalla stortura, dalla vera e propria rottura rispetto all'ordinamento costituzionale della libertà sindacale, della libertà delle rappresentanze professionali, professionali, che è contenuta nel primo comma dell'articolo; ma anche dal comma 2-*bis* che avete voluto a tutti i costi inserire nel testo legislativo. In proposito, vi invito ad un'ultima riflessione. Una norma che prevede che agli uffici di un ente, sia pure ente pubblico, sono destinati i medesimi locali e spazi utilizzati da quell'ente alla alla data di entrata in vigore della legge, e questo in presenza di una sentenza di sfratto, non è una norma di legge, se è vero che nel nostro ordinamento costituzionale la legge deve avere carattere

un provvedimento di legge, è un provvedimento di carattere sostanzialmente giudiziario, contrario a quello adottato dai magistrati. Se così è, qui c'è un vero e proprio conflitto di attribuzione. Stiamo esercitando un potere giudiziario disporre in senso contrario a quello che è stato disposto dalla magistratura in questo caso specifico. Ma noi non abbiamo, per ordinamento costituzionale e civile, questo potere.

che stabilisse che quei locali devono essere liberati. Se era sbagliata quella norma questa lo è molto di più per questa particolarità,

perché si impone all'amministrazione della giustizia un costo aggiuntivo che quella sentenza aveva eliminato; quantomeno, si ricostituisce un rapporto che comporta un onere per l'amministrazione pubblica;

Il 28 ottobre l'Aula del Senato ha approvato una risoluzione con la quale si impegna il Governo a portare in Parlamento, al Senato e alla Camera, la bozza di Piano nazionale delle riforme che deve essere presentata a Bruxelles entro il 12 ottobre.

ebbe a riferire nella seduta dell'altro ieri, da parte della Presidenza del Senato, a calendarizzare anche a partire da martedì pomeriggio la discussione su questo tema. Questi sono i punti, *in primis*, il Governo trasmettesse al Parlamento tempestivamente il deliberato del Consiglio dei Ministri di domani,

eventualmente già discusso in 5a Commissione; infine, che il dibattito si concludesse con la possibilità, entro mercoledì, di

gli schemi legislativi della politica europea non sono stati esaminati negli specifici dettagli, anche perché il presidente Schifani si era impegnato in Aula a concedere alla Commissione il tempo necessario per esaminare tali documenti e per presentare il tutto in Aula entro il 2 dicembre prossimo. Questo è un elemento in più, rafforzativo della necessità che i due passaggi illustrati dal senatore Legnini - sia quello propedeutico, in Commissione, sia quello della discussione in Aula

(abbiamo colloquiato informalmente con il presidente Azzollini, che mi sembra concordi con questo percorso) possiamo dare per acclarato il fatto che entro lunedì avremo il documento e che martedì si avvierà la discussione in Commissione.

alle sue battute finali. Quindi, il nostro Gruppo è favorevole al fatto che tra martedì e mercoledì si proceda esaminando gli argomenti all'ordine del giorno, cioè l'intervento del ministro Maroni, il prosieguo e, mi auguro, la conclusione (anche ai sensi dell'esaurimento dei tempi) della riforma della professione forense e la discussione sulle scadenze europee e sulla mozione Rutelli. Poi, se quest'ultima verrà

solo per ricordarle, nelle more di questo dibattito, che la questione che è stata segnalata dal senatore Legnini e che è stata raccolta anche dal presidente Gasparri riguarda anche e soprattutto la 14ª Commissione,

Non è una questione solo di partigianeria rispetto alla 14ª Commissione, ma o noi approviamo le risoluzioni sull'Europa in quest'Aula, e hanno un seguito, oppure si tratta solo di fuffa europea.

Nell'associarmi alle parole del vice presidente Chiti in occasione della Giornata delle Forze armate, desidero ricordare che oggi alle ore 16, nella nostra Aula, per iniziativa del senatore Marini e della senatrice Bonfrisco, cui ha dato volentieri seguito il presidente Schifani, avrà luogo un concerto di cori alpini in memoria dei caduti in Afghanistan della brigata alpina Julia.

questo è uno dei punti essenziali della riforma. Leggo testualmente l'articolo 25: «1. Sono organi dell'ordine circondariale: *a)* l'assemblea degli iscritti;

Il giudice dipende da chi ha funzioni amministrative e questo determina un conflitto di interessi di cui non possiamo non prendere atto.

assolutamente inconcepibile che l'organo che esercita la giurisdizione, che applica le sanzioni disciplinari, che

dell'avvocatura. È come se il Ministro della giustizia - facendo un parallelo - e il Consiglio superiore della magistratura si unificassero; cosa che non è pensabile perché ciascuno ha delle competenze specifiche, per ragioni molto precise che rispondono anche al principio sulla divisione dei poteri. Quindi richiamo l'attenzione su una norma così delicata, che mette sotto